Grazie

Il Senato è un organo costituzionale e, pertanto, obbligatorio. Deve essere quindi rinnovabile in qualunque momento. settimana scorsa ho segnalato l’impossibilità di procedere al rinnovo del Senato, tenuto conto che le dieci Regioni che hanno due senatori non possono coniugare tutti i requisiti posti dalla Costituzione, ovvero il rispetto dell’equilibrio tra uomini e donne, il fatto che debbano essere attribuiti con un sistema proporzionale, il fatto, ancora più incomprensibile, che i seggi siano attribuiti in ragione dei voti espressi, cioè col metodo proporzionale, e della composizione di ciascun Consiglio, ovvero proporzionale e maggioritario.

il Trentino-Alto Adige, contrariamente a quanto sempre sostenuto (cioè che tale Regione avrebbe espresso due senatori per Trento e due per Bolzano), potrebbe averne non quattro, ma sei.

non sono più state previste le modalità di calcolo dei quozienti elettorali e le modalità di attribuzione dei seggi. Nessuno mi ha dato una risposta e gli interessati mi rispondono che si farà una legge elettorale. Benissimo!

tra i propri membri. prevede che l’ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo. Mi si potrà dire che si tratta di una incompatibilità e che quindi questo consigliere regionale o, meglio, deputato regionale potrebbe dimettersi. Ma nel momento in cui si dimettesse, non potrebbe più fare il senatore!

ho denunciato oggi uno stato dell’arte per cui il Senato non è rinnovabile. Se lei ritiene che fare una comunicazione di questo tipo all’Assemblea sia cosa impropria, allora mi dispiace ma ho sbagliato mestiere, oppure lo ha sbagliato qualcun altro.

la discussione su questo provvedimento ha avuto come oggetto una questione delicata e urgente e, soprattutto, prioritaria. Ci ha imposto un’oculata analisi di tutto il provvedimento che, dopo l’attività svolta in Commissione lavoro, è giunto in Aula. Noi, come opposizione, abbiamo dato il nostro contributo e fatto la nostra parte. L’impianto generale di entrambi i disegni di legge ha rappresentato un tentativo, correggibile su alcuni aspetti, di voler porre fine alla disparità cercando di dare un segnale di equità e dignità al lavoro autonomo e professionale, privilegiando il mondo delle cosiddette partite IVA, liberi professionisti e freelance, rimanendo però esclusi gli im- prenditori. Sappiamo che il mondo del lavoro e l’approccio verso il mercato sono cambiati e stanno cambiando. Le prospettive per chi entra o entrerà nel circuito professionale non sono più quelle di dieci o venti anni fa, ma sono cambiate, ed è giusto che le leggi si adattino a tali cambiamenti. La nostra economia si regge in grandissima parte sul lavoro autonomo, come dimostrato dall’aumento dei lavoratori titolari di partita IVA, i quali però per anni nel mercato del lavoro hanno brancolato nel buio, non vedendosi riconosciuti giusti diritti e garanzie. Uno degli aspetti più interessanti di questo provvedimento è stata la creazione di uno sportello di intermediazione, che raccoglierà le domande e le offerte per il lavoro autonomo e fornirà - almeno così ci auguriamo - le informazioni ai professionisti e alle imprese che ne faranno Occorre però porre in essere le sinergie operative necessarie a far sì che il meccanismo funzioni e non si traduca in un ennesimo sportello contro cui si infrangono le speranze e i sogni di quanti vogliono lavorare. Su questo, come su altri aspetti, abbiamo visto con favore l’approvazione di alcuni nostri emendamenti da parte della Commissione lavoro. Altri poi sono stati recepiti dal relatore che li ha considerati sicuramente un apporto positivo al testo soprattutto al richiamo al tentativo di conciliazione in caso di controversia in ordine al risarcimento dei danni, dello svolgimento delle funzioni che possono e che potevano avere i patronati, i quali, per la loro provata esperienza in campo previdenziale e lavorativo, per la loro presenza capillare sul territorio nazionale, per la loro professionalità e qualificazione, potevano espletare procedure indicate da occorre sottolineare che oggi i centri per l’impiego sono sottodimensionati e hanno bisogno di forza lavoro per garantire quei servizi che noi riteniamo essenziali per le prestazioni. L’estensione della norma agli istituti di patronato avrebbe sicuramente dato più forza e più servizi al mondo del lavoro, ma non è stata possibile; dunque i patronati anche in questo caso rimarranno fuori da questi servizi, pur essendo in molti casi

che, come è noto, è variegato: non esiste solo il lavoro dipendente, ma anche quello autonomo e le partite IVA. È chiaro che a fronte di questo ci saremmo aspettati un intervento molto più determinato e complessivo da parte del Governo. Non è una novità: siamo in fase preelettorale, quindi tutto ciò che accade viene inevitabilmente ricondotto a una logica opportunistica da parte dell’Esecutivo, ma anche messo in sordina da parte dei Gruppi di maggioranza per evitare che, andando ad affrontare seriamente e concretamente temi come quelli del lavoro del lavoro autonomo, si possano avere frizioni all’interno dei Gruppi stessi. Tale atteggiamento ci lascia ovviamente non soddisfatti, perché il taglio del dibattito risulta piegato più all’opportunità e all’opportunismo che invece alla concretezza che dovrebbe caratterizzarne i contenuti. Il relatore ha fatto un buon lavoro, ma non ci ha soddisfatto la reiezione degli emendamenti che abbiamo presentato e che avrebbero dato ulteriore dignità e riconoscimento al lavoro autonomo e soprattutto una reale equiparazione rispetto ai diritti dei lavoratori. Troppo spesso viene dimenticato dal Governo che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non sulla finanza; inoltre, troppo spesso diventa opportunità per finanziare i buchi degli istituti previdenziali piuttosto che per dare una soluzione al futuro pensionistico e previdenziale dei lavoratori.

Ci auguriamo che non ci sia l’ennesimo annuncio slegato dalla concretezza dei fatti, data esclusivamente dal finanziamento delle risorse. delle risorse. Occorre certamente lavorare ancora di più e con determinazione sulla deducibilità delle spese; occorre, senza alcun dubbio, che siano definiti dei livelli, per quanto concerne i professionisti autonomi, riguardo al pagamento delle prestazioni, evitando quel gorgo vizioso per cui alla fine c’è addirittura una sovraesposizione nell’attesa di incassare. Su questo abbiamo fatto dei passi in avanti,

utilizzata in maniera molto strumentale ricorrendo a una lingua straniera per impedire alla gente di realizzare che si trattava di una riforma del lavoro. Allora il Governo scelse - e la maggioranza ovviamente si piegò - di tenere distinto il lavoro autonomo dal lavoro dipendente.

quelle svolte positive di cui ci sarebbe invece bisogno. A fronte di ciò, il nostro sarà un voto di astensione, valutando in futuro, con l’attuazione del provvedimento stesso, che cosa ne deriverà e se saremo di fronte all’ennesima boutade preelettorale. Siamo di fronte ad una riforma costituzionale che il Governo sta cercando di imporre con metodi che nulla hanno a che fare con il rispetto della democrazia, ma che tutto hanno a che fare con sistemi di propaganda da venditori di detersivo,

Sacconi che ha portato avanti un provvedimento che oggi verrà posto in votazione e che è estremamente interessante e lungamente atteso, poiché riguarda disposizioni importanti per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale ed è rivolto a tutta le attività professionali e ai freelance. Il primo punto qualificante di questo disegno di legge è quello di riconoscere finalmente la dignità Grazie rappresentanti di questo importante tessuto economico del nostro Paese, che sono i liberi professionisti, avanzavano già da tempo.

che, come sappiamo, molto spesso si caratterizzano - ahimè - per tempi di pagamento enormemente lunghi (in alcune Regioni tali

di discussioni al nostro interno: si dispone la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la formazione e l’aggiornamento professionale ancorché entro il limite di 10.000 euro l’anno, nonché le spese di iscrizione a convegni o congressi. Inoltre, vale la pena di ricordare come siano altresì deducibili integralmente, entro il limite di 5.000 euro l’anno, le spese sostenute dal lavoratore autonomo per i servizi di certificazione delle competenze, orientamento e ricerca. è lo sportello dedicato al lavoro autonomo. Innovativa e interessante è la previsione di cui all’articolo 9 secondo cui i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni con gli ordini professionali. sull’accesso agli appalti pubblici. Si tratta di una disposizione che ritroviamo nell’articolo 11; tale disposizione è tesa a consentire che i lavoratori autonomi possano partecipare agli appalti pubblici e favorisce l’accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche. Bisognerà comunque coordinare questa disposizione con il decreto del Governo sugli appalti pubblici che non annovera i liberi professionisti nell’elenco dei soggetti che rientrano nel concetto di nel concetto di «operatore economico» ammesso a partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Per quanto riguarda l’accesso ai fondi europei, ai fini dell’accesso ai fondi strutturali, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese. Si tratta di una norma importante perché consente ai liberi professionisti italiani di poter finalmente partecipare ai bandi europei, proiettandoli in una dimensione transnazionale, né più né meno di quanto succede negli altri Paesi.

parentale da tre a sei mesi entro i tre anni di vita del bambino. Per quanto concerne gravidanza, malattia e infortunio si introducono disposizioni di notevole impatto, poiché è previsto che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori che prestano che prestano la propria attività in maniera continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, ma la sua esecuzione rimane sospesa senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare. Interessante ci sembra poi la possibilità

al lavoro da un familiare della lavoratrice stessa, o anche da eventuali soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza. Questo sarà un ambito certamente tutto da esplorare che potrebbe riservare delle sorprese positive.

indispensabile. Allo stesso modo è importante e va nel segno dell’equità l’equiparare alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Anche se forse sarebbe il caso il caso di non fermarsi alle sole malattie oncologiche e di estendere la previsione anche alle altre. In Commissione tuttavia questo articolo è stato soppresso e questo per noi è un vero peccato. Per quanto concerne le previsioni riguardanti il lavoro agile, si tratta di una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, di un nuovo strumento

laddove sono sempre più diffuse figure professionali ibride, che stanno a metà tra la ricerca e la gestione del cambiamento nei processi organizzativi e produttivi, realizzando una piena integrazione tra lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione. Le parti possono accordarsi sul luogo di lavoro, che può essere in parte all’interno dell’azienda e in parte fuori, così come l’orario di lavoro è privo di vincoli rigidi. Importante, per una piena chiarezza delle norme che presiedono al lavoro agile, è l’aver previsto riguardo al trattamento giuridico che il lavoratore impegnato nel lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante al lavoratore che svolge le medesime Grazie di accordarsi liberamente per adattare le regole del rapporto di lavoro che intendono intraprendere alle loro esigenze concrete, compresi orari e luoghi di lavoro, in modo da mettere insieme le esigenze variabili degli obiettivi da raggiungere nella produzione con le esigenze personali o gli stili di vita del lavoratore. Quindi, al netto di alcune criticità

Signor Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, colleghe e colleghi, in questi ultimi anni, a seguito anche dell’affermarsi delle nuove tecnologie e della globalizzazione dei mercati, si è assistito a profondi mutamenti nel sistema produttivo e con esso anche in quello organizzativo del lavoro. Sempre di più il lavoro diventa flessibile e non è più caratterizzato dal posto fisso per la vita, da un unico luogo di lavoro e neppure da un orario fisso. Sempre di più i lavoratori svolgono la loro attività in forma non solo autonoma, ma anche e soprattutto tramite tipologie di contratto «atipiche». Purtroppo proprio queste forme atipiche hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, andando a costituire nel mondo del che più di altre rischia di scivolare verso la povertà e verso l’insicurezza della continuità lavorativa e, dunque, anche nella pianificazione della propria vita

che ogni individuo si possa personalizzare il proprio lavoro sia in base alla possibilità di esprimersi e realizzarsi, sia in base alle proprie esigenze logistiche e di orario. Questa - con le dovute tutele e la dovuta sicurezza - è una buona espressione del mondo moderno del lavoro. Dunque, mentre la flessibilità assume sempre più un criterio dominante nell’organizzazione del lavoro di oggi, è estremamente importante garantire anche sicurezza al lavoratore. Il provvedimento che stiamo per approvare in Aula oggi è espressione di politiche mirate che devono appunto servire a migliorare la situazione delle categorie che sono particolarmente e e criticamente esposte (dal punto di vista del fisco e nel modo di pensare della gente), a cominciare da quelle che non fanno riferimento a uno specifico albo professionale. Questa legge riguarda soprattutto i giovani, le generazioni impiegate nelle nuove professioni dei servizi e del terziario di ultima generazione. L’obiettivo è quello di perseguire l’universalità delle tutele dei lavoratori autonomi, e questo testo sicuramente è un passo verso la giusta direzione. Certo, non è risolutivo delle difficoltà di un settore così vasto e particolarmente eterogeneo e articolato, tuttavia le novità introdotte ci convincono soprattutto nella parte relativa al lavoro da casa o da remoto, che ha l’obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro, andando incontro a modelli che guardino sempre più all’efficienza e ai risultati. Un plauso, dunque, alle modifiche introdotte come l’estensione del congedo parentale anche ai padri iscritti alla gestione separata, e, per entrambi i genitori, il periodo di fruizione ampliato da tre a sei mesi e dal primo al terzo anno di vita del bambino, nonché l’esclusione dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo dei rimborsi delle spese di alloggio e vitto relativi alle trasferte in seguito a un incarico conferito dal committente e l’estensione delle politiche attive anche ai lavoratori autonomi con i centri per l’impiego che dovranno dotarsi di sportelli dedicati. Lasciatemi, però, esprimere qualche riflessione e, tuttavia, anche qualche giudizio molto critico - lo sottolineo - nei confronti della mancata volontà di accettare qualunque modifica e semplificazione, anche logica, su alcune principali misure che avrebbero potuto apportare delle migliorie in ambito di semplificazione senza, tra l’altro, introdurre maggiori oneri per lo Stato. Il comma 1 dell’articolo 19 concerne la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, 2016 formativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Ritengo del tutto inutile presentare l’informativa tutti gli anni qualora non ci siano modifiche; sarebbe stato più semplice e anche più efficace che questo tipo di informativa avvenisse nel momento in cui vi siano dei cambiamenti. modo, sono dell’avviso che andrebbe approfondita la materia della gestione separata INPS entro la quale ricadono categorie molto diverse tra loro (dai professionisti non iscritti a un albo professionale ai collaboratori subordinati, agli amministratori di società). È necessario andare incontro a una riorganizzazione del settore, prevedendo forme diversificate di gestione separata. Un altro emendamento proposto, ma che, purtroppo, non ha avuto l’attenzione da parte del Governo,

per le trasferte di lavoro, in particolare alle forme con cui esse concorrono a formare il reddito. Dobbiamo stare attenti a creare un provvedimento che diminuisca la burocrazia e non ne produca di nuova; un provvedimento che crei certezze del diritto e non che aggiunga altre incertezze. Permettetemi di sollecitare la vostra attenzione anche su un altro aspetto che sicuramente esula da questo provvedimento, ma che è da considerare pur sempre un intervento a favore dell’imprenditoria e del lavoro autonomo in un’accezione più estesa. Penso sia necessario e importante riflettere su una revisione del sistema previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, alla luce del fatto che i contributi pagati per questa categoria sono superiori a quelli pagati da qualunque altra categoria di lavoratori. Auspico che presto venga riequilibrata la contribuzione previdenziale tra lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e quella versata da altre categorie, attraverso l’eliminazione della doppia contribuzione nel caso in cui i contributi vengano pagati doppi, sia per lavoro dipendente sia per la gestione separata, e attraverso la ricongiunzione non onerosa dei vari periodi contributivi. Bisogna dire che il disegno

Siamo però convinti che la strada intrapresa sia quella giusta e che le riforme quelle già avviate e quelle preannunziate - vadano sostenute, approvate e attuate. Signor Presidente, signor Sottosegretario,

saluto gli studenti e i docenti dell’Istituto di istruzione superiore «Piaget-Diaz» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

È vero che anche la collaborazione coordinata e continuativa costituisce lavoro autonomo, perché il soggetto può organizzarsi con mezzi propri, tuttavia si tratta di una fattispecie in concreto molto diversa. nel contratto d’opera vero (cioè il lavoro autonomo) la prestazione lavorativa è unica e questa è la vera differenza con ogni altra forma di contratto. Per ottenere un altro prodotto e un servizio diverso da quello inizialmente richiesto, bisogna fare un altro contratto. Il prestatore d’opera vero è colui che tratta con un pubblico ampio e differenziato, con il quale conclude molti contratti d’opera, mentre il collaboratore coordinato e continuativo, visto il maggior impegno temporale di questo tipo di rapporto, avrà pochi clienti committenti (spesso uno solo o uno principale), con la conseguenza che, di fatto, la sua sopravvivenza economica e professionale finirà con il dipendere dai suoi pochi committenti, che daranno direttive sempre più vincolanti. Quindi, di quale autonomia parliamo? Non si capisce. Se lo dobbiamo dire in italiano, questo è lavoro parasubordinato. Ecco il pericolo.

inoltre ogni responsabilità al datore di lavoro sul tema della sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro non avrà più alcuna responsabilità verso i lavoratori:

in tutto questo, si toglie ogni vincolo al datore di lavoro, ma si chiede una cosa molto importante. Il famoso controllo a distanza,

il mercato del lavoro nei Paesi occidentali e in Italia è coinvolto da almeno trent’anni in un profondo processo di trasformazione. Si tratta di un mutamento estremamente veloce e instabile, incapace di essere catturato da leggi e regolazioni amministrative, che risultano velocemente obsolete quando eccessivamente dettagliate, oppure sostanzialmente inefficaci quando troppo generiche. La rapidità delle trasformazioni in atto ha ragioni demografiche, sociali, politiche ed economiche complesse; è però l’innovazione tecnologica ad essere individuata dalle istituzioni internazionali e dalla dottrina come il principale fattore di cambiamento del mercato dei lavoro, almeno nel breve termine. In questo contesto mutevole, sono convinto che una formazione adeguata dei lavoratori (non solo di quelli nuovi) sia possibile solo superando i dogmi della linearità e della separazione che affliggono la scuola e la formazione continua italiana. È necessario più lavoro durante la formazione iniziale (alternanza e apprendistato) e più formazione di qualità durante il lavoro poi (formazione continua); allo stesso modo, per formare le soft skill sempre più richieste dalla società della conoscenza, è importante tornare a credere nella valenza formativa ed educativa del lavoro e integrare sapere teorico e sapere pratico, superando la diffusa gerarchizzazione dei canali formativi. Convinti interventi in materia di istruzione e formazione primaria, secondaria e terziaria, anche nell’ottica di incrementare l’offerta formativa nei settori ad alta specializzazione tecnologica, appaiono più efficaci di misure di riqualificazione costante gestite dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive Queste sono certamente importanti per la gestione emergenziale di lavoratori in esubero e disoccupati, ma da sole non determinano quel cambio di paradigma di cui ha bisogno l’intero sistema formativo italiano. Di fronte ad un simile panorama, uno degli obiettivi principali che si è posto il legislatore è stato quello di costruire per le imprese e i lavoratori un quadro normativo di semplificazione e di snellimento burocratico e di valorizzare l’innovazione tecnologica e le competenze acquisite, per affrontare una vera e propria sfida dell’occupazione in una diversa concezione del mercato del lavoro. Cambiano i modelli organizzativi della produzione, ma cambia anche il modo di concepire il lavoro, in questa quarta rivoluzione industriale di cui nessuno può prevedere con certezza la dimensione e il relativo passo. La nostra sola certezza è che viene meno un vecchio mondo, impostato su gerarchie verticali e sulla mera esecuzione seriale delle direttive impartite.

La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono ormai più visti in negativo, ma anzi rappresentano un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. È quindi evidente che il prestatore di lavoro del presente e del futuro possa arrivare a svolgere la propria opera all’interno di un progetto, una missione, un incarico, una fase dell’attività produttiva. È in questa direzione che si orienta il jobs act dei lavoratori autonomi: un ripensamento del lavoro in un’ottica più intelligente, con una messa in discussione dei tradizionali vincoli legati a luoghi e orario, e a una maggiore responsabilizzazione quanto ai risultati; una misura che, a mio avviso, può incentivare realmente lo smart working in un’ottica di crescita profes- sionale del lavoratore e di miglioramento della competitività per l’impresa. Il provvedimento affianca politiche mirate a supporto delle esigenze della donna multitasking, che sempre più spesso si trova a dover conciliare ruoli plurimi tra casa, famiglia, lavoro e cura di genitori anziani. Previo accordo tra le parti, si definiscono forme di organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi, senza vincoli di orario o luogo di lavoro, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La mansione può essere eseguita in parte all’interno dell’azienda e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Lo smart working non è quindi una tipologia contrattuale, perché tutte le tipologie contrattuali possono realizzarsi con modalità agili, ma ben si adatta ad una logica di tipo orizzontale, che lascia spazio alla creatività e alla responsabilità. L’agilità della prestazione lavorativa diventa quindi un concetto che supera, pur rimanendo ad essa funzionale, la mera esigenza di garantire una migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia. Grazie a questo provvedimento, tra le altre cose, i liberi professionisti saranno in primo luogo tutelati, perché si proibisce all’impresa di instaurare eccessive sproporzioni fra diritti e obblighi, superando l’abuso di dipendenza economica dell’articolo 9 della legge n. 192 del 1998. È inoltre di tutta evidenza che deve essere organizzato anche un efficace programma di welfare per i professionisti, soprattutto per i più giovani, per agevolare loro l’ingresso nel mondo professionale, ma anche in riferimento alle ulteriori fasi di vita lavorativa che coinvolgono i colleghi più anziani. È proprio in questa direzione che dobbiamo leggere le norme contenute nel cosiddetto statuto dei lavoratori autonomi: azioni positive rivolte al sostegno della genitorialità, al sostegno del reddito e al supporto dell’evoluzione tecnologica necessaria per l’espletamento dell’attività professionale. Abbiamo affrontato in questo provvedimento anche il tema dei congedi parentali: le nuove norme elevano il limite di durata, da tre a sei mesi, dei trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori e abbiamo esteso il diritto al suddetto trattamento economico con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino. Anche in tema di indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS abbiamo esteso il diritto

Sempre in tema di welfare per i lavoratori “agili”, considerato che la loro prestazione risulta maggiormente fluida e flessibile, e prevede una maggiore autonomia del dipendente rispetto ai propri orari di lavoro, abbiamo introdotto il cosiddetto «diritto alla disconnessione», che si configura come strumento utile per il passaggio ad una nuova concezione del lavoro, valutate anche le necessità di riposo dei lavoratori. Esso, infatti, non si pone come un mero divieto: all’articolo 16 del provvedimento si parla di: «misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione» e si configura, quindi, come un impegno nella ricerca di soluzioni ottimali perché la disconnessione sia garantita. Non è un caso che la predisposizione delle concrete risposte alla necessità di disconnessione siano lasciate, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alle parti più vicine all’organizzazione del lavoro, ossia all’accordo individuale. Ritornando sul tema della formazione, poi (cui accennavo in premessa), ribadisco la necessità di predisporre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale attraverso l’utilizzo dei fondi interprofessionali: questo è un ingrediente fondamentale per il lavoro del futuro e per il lavoro agile. Mi accingo a concludere: noi, come legislatori, riteniamo che il cosiddetto statuto dei lavoratori autonomi possa garantire un sistema di tutele e di welfare finora non riconosciuto a questa categoria di lavoratori. Pensiamo che questa sia la strada giusta da prendere: è un percorso di equità e necessità, per favorire e non svilire le intelligenze vivaci del nostro Paese e per rimanere al passo con i continui cambiamenti che la società impone al mercato del lavoro. È per questi motivi che il Gruppo di Area Popolare voterà convintamene a favore di questo provvedimento, nell’auspicio che si possa pervenire quanto prima alla sua approvazione definitiva.

debba essere tutelato in tutte le sue forme, soprattutto quando si tratta di piccole e medie imprese. Quindi bisogna spingere affinché lo Stato crei un ordinamento che consenta all’imprenditore di poter fare impresa senza avere lacci burocratici inutili. Non da meno, lo Stato deve individuare, attraverso lo studio del momento storico, le esigenze del piccolo imprenditore. Questo provvedimento è scisso, suddiviso in due: da un lato c’è quello che stiamo dicendo in questo momento, e cioè una regolazione che opera direttamente sul lavoro autonomo, ma dall’altro vi

perché dell’articolo 1 all’articolo 14 contiene norme che, anche a nostro avviso, tutelano maggiormente il lavoro autonomo non imprenditoriale.

lavoro autonomo non imprenditoriale che devono essere regolate. Bisogna dunque assolutamente fornire tutele. Ovviamente, sto parlando non soltanto di tutele in ambito civile, ma di tutele anche in ambito previdenziale. Orbene, in ambito civile il provvedimento ha effettivamente qualcosa di buono. In particolare, faccio riferimento al

potrebbe magari anche essere qualcosa all’ordine del giorno (anche se non dovrebbe esserlo, è più comprensibile perché, magari, si è tutti in crisi). Ma non è comprensibile quando la pubblica amministrazione ritarda il pagamento dei professionisti: questo è inaccettabile. E su queste forme

quindi ovviamente anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi non imprenditori come nel caso di specie, il Movimento 5 Stelle c’è. Effettivamente, abbiamo dato il nostro appoggio a quelle norme riguardanti l’introduzione di regole più robuste per sanzionare anche le pubbliche amministrazioni che ritardano il pagamento di questa tipologia di lavoratori. Altro punto molto interessante del provvedimento sono le tutele nel caso di modifiche unilaterali da parte del committente. Questo è un aspetto importante perché, molto spesso, questo tipo di lavoratori autonomi non sono tutelati allorquando il committente inserisce anche all’interno del contratto alcune clausole che possiamo definire, in realtà, anche vessatorie. Bisogna lavorare, però, e molto spesso il lavoratore autonomo accetta comunque. In questo caso abbiamo voluto inserire l’annullabilità di quel contratto che prevede alcune clausole che vanno a attaccare il lavoratore autonomo. Faccio particolare riferimento alle tutele in caso di recesso senza un congruo preavviso e alle modifiche unilaterali del contratto. Altro punto positivo è una maggiore tutela per l’attività inventiva. Questo è un punto fondamentale. Poi c’è la parte relativa alla semplificazione, che ci sta molto a cuore, come dicevo inizialmente. Bisogna assolutamente semplificare, perché uno Stato poggiato sulla burocrazia è uno Stato che dà da mangiare anche, purtroppo, al malaffare: tanta burocrazia, tanto malaffare; poca burocrazia, poco malaffare.

la possibilità di creare strumenti per la deflazione del contenzioso (fino a qui potrebbe anche essere

veramente libero di denunciare il datore di lavoro. Diversamente non ci saranno più strumenti di controllo. E, quindi, “marameo” alla vigilanza sul lavoro.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, preliminarmente voglio ricordare che questo provvedimento è il secondo intervento che si muove nella logica della riforma del mondo del lavoro. Per il lavoro dipendente il Governo ha proposto il cosiddetto jobs act

Occuparsi di questa riforma è necessario per non ampliare le disparità dei diritti tra chi ha un “posto fisso” e chi, nel settore privato, ogni giorno deve fare i conti con stipendi di livello mediamente più bassi di quelli pubblici e con il rischio di non vedersi rinnovato il contratto. La saga dei furbetti del cartellino, intanto, si arricchisce ogni giorno di nuovi episodi, ultimo della serie quello del Comune di Sulmona. E questo episodio mi porta a fare due riflessioni. fare due riflessioni. Innanzitutto, i provvedimenti punitivi, anche momentanei, necessitano di norme ancora più concrete in tal senso. La seconda riflessione è che l’assenza di lavoratori pubblici dal posto di lavoro evidenzia - secondo me - la presenza di piante organiche ancora troppo ampie e, quindi, la necessità di un’ulteriore semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione che consenta di snellire gli organici. Detto questo, il disegno di legge del Governo si inserisce in quella riforma generale del mondo del lavoro di cui abbiamo detto prima. Noi riteniamo che il lavoro autonomo debba avere delle forme proprie che non possano essere assimilate a quelle del lavoro dipendente. Non si può, inoltre, far finta che negli ultimi trent’anni il mondo del lavoro non sia cambiato a livello globale e che ciò non condizioni anche i modelli da adottare nel nostro Paese. bisogna certamente definire un quadro di regole, di disposizioni, per fornire risposte concrete a questo ampio mondo produttivo rappresentato dai lavoratori autonomi. Rimane, comunque, una evidente disparità, difficile da colmare, tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, rispetto ai redditi e ai diritti: il diritto di ammalarsi, di sostenere le cure della propria famiglia e la copertura continuativa dei periodi di contribuzione ai fini previdenziali. L’augurio è che l’apposita delega introdotta dalla Commissione tenga conto di tutti i rilievi e delle problematiche in tal senso emerse durante il dibattito. Noi, consci delle problematiche che affrontano ogni giorno i lavoratori autonomi, avevamo proposto una serie di emendamenti tesi a ridurre tale divario.

parentale rispetto ai diritti delle lavoratrici autonome contemplate nel disegno di legge oggi in discussione. Vi è poi la possibilità di dedurre i costi di formazione ai fini IRPEF, che fa pensare a una idea di lavoratori in continua specializzazione e, quindi, fa ipotizzare disposizioni adatte ai più giovani, ai ragazzi che iniziano una carriera lavorativa, ma sicuramente utili anche per persone che decidano di cambiare attività lavorativa. Nell’attuale assetto normativo si sono già registrati diversi casi di applicazione di questa forma di flessibilità, sulla base di iniziative aziendali con i singoli lavoratori oppure in forma collettiva attraverso specifiche inte Peraltro, un primo riferimento è già stato introdotto con l’articolo 2 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 sulla detassazione dei premi dove, incidentalmente, si chiarisce che, per lavoro agile, deve intendersi una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Così, nel solco tracciato e sulla scorta delle esperienze della contrattazione collettiva, si può dire che lo smart working rappresenta non una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità diversa di esecuzione della normale prestazione, senza imporre uno specifico luogo di lavoro. Il lavoro agile si differenzia anche dal telelavoro; in quest’ultimo caso, infatti, il datore di lavoro è tenuto a porre a disposizione del dipendente una postazione di lavoro fissa ove questi sarà tenuto a svolgere l’attività assegnata.

Lo smart working è appunto un’opportunità di risparmio per le imprese: oltre alle agevolazioni previste in tema di detassazione, con questa modalità di esecuzione della prestazione si possono infatti escludere le indennità legate a trasferte e alle missioni, in quanto non si presuppone la presenza fisica presso la sede di lavoro, e riferite al temporaneo allontanamento da essa. Rimangono aperti, tuttavia, due temi che nell’attuale assetto normativo potrebbero generare incertezza: e l’eventuale infortunio in itinere; tema, quest’ultimo, che il testo per la prima volta intende regolare. Importante è l’introduzione del diritto alla disconnessione, per scongiurare il rischio che il lavoratore diventi schiavo della connessione permanente. Diverse grandi aziende tedesche e francesi hanno già raggiunto accordi per evitare il fenomeno del cosiddetto e oltralpe si sta discutendo di inserire il diritto alla disconnessione nell’ordinamento. Il tema è quindi tanto attuale quanto delicato e non può essere lasciato alla improvvisazione. Oggi questa modalità di lavoro ha un interesse crescente nelle aziende: il 17 per cento delle grandi imprese italiane ha avviato nel 2015 progetti progetti organici di smart working (erano l’8 per cento nel 2014), introducendo in modo strutturato nuovi strumenti digitali, policy organizzative, comporta- menti manageriali e nuovi layout fisici degli spazi. A ciò si aggiunge il 14 per cento di grandi imprese che si dichiara intenzionato ad avviare progetti e un ulteriore 17 per cento che ha avviato iniziative per particolari profili, ruoli o esigenze del personale. Quasi una grande impresa su due sta andando in modo strutturato o informale verso il nuovo approccio all’organizzazione del lavoro; sono molte le aziende che in Italia hanno già progetti di smart working in corso. Sicuramente questo provvedimento intraprende un percorso al passo con i tempi. Va rilevato, però, che una riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale avrebbe richiesto ulteriore forme di investimento da parte dello Stato. Al contrario, il disegno di legge in esame mette in campo pochissime risorse economiche, tra l’altro distogliendole da fondi e capitoli di spesa già dedicati al mondo del lavoro.

La nostra idea, comunque, è ritenere che la vera riforma del lavoro privato vada fatta innanzitutto affrontando il tema della fiscalità che grava su chi lavora, a partire dal livello dalle aliquote, per passare al modello delle deduzioni e detrazioni fiscali dall’imponibile IRPEF. Oggi in Italia il dipendente gode di detrazioni fiscali da lavoro molto più ampie di quelle di cui può beneficiare un lavoratore autonomo, perché si considera ancora il lavoratore autonomo un potenziale evasore. Va invertito questo tipo di logica, ponendo il lavoratore autonomo in condizione di godere di una detrazione fiscale da lavoro maggiore rispetto a quella prevista per il lavoratore dipendente, in modo da consentirgli di pagare le imposte solo sulla parte effettivamente non necessaria al proprio sostentamento. Il Gruppo Forza Italia esprimerà voto favorevole sul disegno di legge perché, anche se questo provvedimento non ci soddisfa in pieno, rappresenta, certamente, un primo importante passo verso il riconoscimento di questa categoria di lavoratori autonomi.

Nello stesso disegno di legge si affronta il tema del lavoro agile e di come il lavoro debba cambiare in base ai mutamenti della tecnologia con l’obiettivo di conciliare tempi di vita e di lavoro con la produttività: tutto in uno stesso provvedimento, per rendere il nostro Paese moderno ed efficiente, con più diritti e con un welfare in grado di sostenere il futuro delle prossime generazioni e delle nostre imprese.

Ricordo che, quando il 9 aprile 2014 arrivò in Parlamento la delega sul lavoro, il jobs act, uno degli impegni che abbiamo assunto è stato quello di tracciare una linea di demarcazione tra il lavoro subordinato e il lavoro parasubordinato e autonomo. Con il decreto attuativo della legge delega n. 81 del 2015 è stato chiarito che ogni rapporto di lavoro, ancorché di natura parasubordinata e autonoma, che si concretizzi in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità siano organizzate dal committente anche con riferimento

e, dall’altro lato, anche in questo provvedimento si definisce in maniera chiara il lavoro autonomo come lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Questo confine - lo ricordava ieri anche il Sottosegretario - è stato una delle fondamenta della riforma del lavoro, contenuta quindi sia nel jobs act che nel jobs act del lavoro autonomo, per smascherare abusi e false par- tite IVA. Senatore Barozzino, quante volte abbiamo parlato in quest’Aula delle false partite IVA e della necessità di porre un confine rispetto al lavoro autonomo e al lavoro dipendente? Quante volte l’opinione pubblica si è interrogata su questi temi? Ecco, noi li abbiamo affrontati e abbiamo

La sfida quindi che oggi siamo chiamati ad affrontare è assicurare tutele, strumenti di assistenza e sostegno a quei lavoratori e a quelle lavoratrici. Sono stati molto puntuali gli interventi del mio Gruppo, che hanno ricordato le principali tutele. Ne ripercorro solo alcune: si affronta il tema della formazione con il rafforzamento delle deduzioni delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, stabilendo che la formazione

clausole abusive, della maternità e del congedo parentale. Potranno avvalersi del congedo parentale sia le mamme che i papà nel limite complessivo di sei mesi nell’arco di vita dei tre anni Si avrà la possibilità di ricevere l’indennità di maternità pur continuando a lavorare e, in caso di malattia o infortuni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per questi lavoratori è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio. I liberi

Il lavoro agile è definito come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Invito chi critica tale tema a uscire da queste stanze e capire dove sta la realtà, cosa succede, quanti accordi ci sono già sul lavoro agile, perché il mondo va avanti. E va chiarito che stiamo introducendo non una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario e di luogo di lavoro.

Noi avremo aziende organizzate per processi, per risultati e solo quindi importanti modalità di lavoro diverse. Con questo disegno di legge il lavoro agile viene incoraggiato. C’è un’altra disposizione legislativa che è contenuta nella legge di stabilità dell’anno scorso e che quest’anno il Governo rafforzerà:

È per questo che il testo del Governo, come si è presentato al Parlamento, raggiunge un punto di equilibrio, che la Commissione ha confermato nella proposta del testo per l’Assemblea.

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione del corso di diritto pubblico comparato attivato presso l’Università degli studi di Perugia, che sta assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

prevede la trattazione delle mozioni sui tumori femminili e sul rinnovo dei contratti delle Forze di polizia. Nella seduta pomeridiana alle ore 16,30, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata alle ore 15 di martedì.

Presidente, mi trovo nella strana condizione di dovere operare “la scelta di Sophie”. Infatti, da Presidente della Commissione ambiente sottolineo che la Commissione ha lavorato a lungo - e credo proficuamente - per arrivare a un testo peraltro ampiamente condiviso. A tal proposito, voglio ricordare a questa che su questo tema si era espressa perché - se non ricordo male - già nel 2013, proprio su richiesta di un parlamentare del Gruppo di Forza Italia, era stata dichiarata l’urgenza del provvedimento e addirittura si paventava l’ipotesi che il provvedimento stesso potesse arrivare in Aula saltando il passaggio in Commissione. D’altro canto, mi trovo nelle condizioni di essere il primo firmatario

Questo è un tema fondamentale, che riguarda e interessa non soltanto gli schemi idrici (quindi gli interessi del comparto agricolo, per altro di primaria importanza nel nostro Paese),

che il Ministero, nel proprio apparato burocratico e - ahimè - anche nella guida politica, intendeva cambiare il vertice della gestione commissariale, tanto che aveva proposto un precedente atto di sospensione e sostituzione del commissario, salvo poi dimostrarsi che tale atto era infondato e assolutamente illegittimo. In quel momento si preferì buttare

ma anche dai risultati gestionali che si erano raggiunti in termini di capacità di spesa e di efficacia ed efficienza della spesa

arrivati a sopprimere delle linee di intervento che erano assolutamente positive e che producevano effetti di tutela e promozione delle DOP e del marchio Italia in genere.

Siamo nel 2016 e abbiamo 136 procedure di infrazione comunitaria. Possiamo, quindi dire che una gestione quantomeno dissennata e non attenta ha prodotto danni piuttosto gravi. I consorzi hanno delle funzioni molto importanti perché, oltre a garantire la parte irrigua, devono garantire anche la bonifica

il numero degli operai, perché i consorzi, insieme alle comunità montane, sono gli ultimi enti che hanno ancora gli operai idraulici che intervengono sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua

Presidente, questo argomento meriterebbe una discussione in un’Aula piena e molto attenta, perché stiamo parlando di uno degli elementi essenziali per la vita: l’acqua La nostra mozione ha come obiettivo quello di chiedere un impegno veramente straordinario da parte del Governo affinché venga avviato un monitoraggio completo delle opere necessarie alla rete infrastrutturale idrica, segnalando, in particolare, le opere avviate e non completate, in maniera tale da avere un censimento preciso di ciò che si è incominciato e e che purtroppo non si è ancora concluso. Occorre agire attraverso un coordinamento strettissimo

attraverso un incremento della dotazione disponibile per la programmazione 2014-2020, adesso vi sono almeno 800 milioni di euro a disposizione per interventi immediati a favore della gestione del piano irriguo nazionale e quindi per interventi che devono essere orientati, come prima dicevo, soprattutto ad azioni di completamento della rete. a dare priorità, in questa spesa, agli interventi che riguardano il Mezzogiorno d’Italia e le isole, dove vi

«ad integrare l’implementazione del risparmio idrico tra i criteri centrali degli interventi». a procedere a una riorganizzazione del sistema dei consorzi di bonifica, che in qualche caso non sono un buon esempio di amministrazione e diventano, diventano, invece, una sede di difficile gestione di un bene comune di assoluto rilievo come l’acqua e, soprattutto, l’acqua Dobbiamo stare molto attenti alla combinazione virtuosa del multisettoriale Non è pensabile che abbiamo ancora in molte città le reti acquedottistiche piene di falle, che continuano a sprecare una quantità impressionante di risorsa idrica,

gli eventi che ci accompagnano, purtroppo, in ogni autunno e primavera, quando arrivano le cosiddette bombe d’acqua, fenomeni così devastanti che sono frutto della mutazione del sistema climatico globale e del cambiamento del clima

delle nostre popolazioni e per contribuire alla rinascita economica del Paese. L’acqua è un bene essenziale anche in questa prospettiva. Questi sono gli obiettivi della nostra mozione, che poniamo all’attenzione del Governo.

ci costringa tutti ad un supplemento di responsabilità. Non credo davvero sia il momento per i giochi d’Aula e non ritengo davvero accettabile che soltanto per verificare una

per il lavoro che ci attende nelle prossime settimane, che in un momento in cui i cittadini italiani guardano con particolare attenzione a ciò che il Parlamento vorrà e saprà fare, e considerata

XVII) Signor Presidente, colleghi, l’argomento proposto dalle mozioni al nostro esame assume grande importanza per l’ammodernamento delle reti irrigue, in particolare nel Sud del nostro Paese, e per la contestuale attenzione richiesta nell’utilizzo della risorsa acqua. In questo ambito molti sono gli aspetti critici e le mozioni hanno il merito di individuarne alcuni: l’invecchiamento delle strutture, la mancanza di ristrutturazione e ammodernamenti, l’incompletezza di molti schemi idrici, la sempre più evidente difficoltà economica, finanziaria e operativa della maggior parte dei consorzi di bonifica, soggetti attuatori di eventuali investimenti. Argomenti molto vasti e cruciali, sui quali però non mi soffermo. Intendo invece sottolineare la necessità di integrazione delle mozioni con alcuni elementi che ritengo altrettanto fondamentali e che si riassumono nell’esigenza di implementare in modo ripetuto azioni di efficienza nelle iniziative di infrastrutturazione del Paese, attraverso l’adozione di una imprescindibile prospettiva di sistema. Il primo punto è questo. Le esigenze di ammodernamento in parte legate ai cambiamenti climatici che le stesse mozioni evidenziano devono vedere una contestuale azione di efficientamento: efficienza nell’uso delle risorse idriche che permetta l’indispensabile ottimizzazione del quoziente volume utilizzato-superficie irrigata a mezzo dell’adozione di tecnologie avanzate, sia attraverso azioni sull’hardware (dimensionamenti e distribuzione) sia per la parte software (metodiche di gestione supportate da tecnologie smart); efficienza energetica in special modo per le reti caratterizzate da sollevamento meccanico delle acque e, quindi, da ingenti consumi energetici. I due precedenti argomenti dovrebbero rappresentare uno standard, sia per i progetti in corso sia per quelli di futura attuazione, divenendo un vero e proprio valore aggiunto, anche in relazione agli impegni che il nostro Paese ha assunto lo scorso anno a Parigi, va assumendo nell’ambito del pacchetto europeo dell’energia e sta per assumere

Vi è poi un altro elemento. In merito al bilancio idrico delegato, al prelievo idrico dal corso d’acqua, all’accumulo in volumi di invaso e alla successiva consegna ai punti di prelievo previa misurazione, si ritiene necessario il coinvolgimento dei distretti idrografici, cui la normativa di settore demanda compiti specifici sull’equilibrio del bilancio medesimo. Allo stesso tempo, si ritiene necessario uno specifico impegno legato alla ricognizione dei volumi disponibili nei bacini di accumulo delle dighe, anche in relazione all’effettivo utilizzo delle medesime, sia per ragioni di progressivo interramento, sia per ragioni legate ad eventuali limiti di invaso all’esercizio delle strutture. In conclusione, in merito al programma mini idroelettrico, che una mozione in particolare cita che si condivide pienamente quale azione di recupero di energia altrimenti dissipate, si ritiene necessario l’impegno del Governo per un’azione forte e chiara per la produzione su tutte le reti, in pressione o no, esistenti o in progetto. E si prevede l’approvazione di percorsi percorsi amministrativi dedicati e semplificati di intesa con le Regioni, con l’obiettivo di raggiungere la sostenibilità economica di questo tipo di applicazione ad impatto nullo,

sulle infrastrutture irrigue e sull’utilizzo delle risorse idriche siano assolutamente prioritari. Il Governo, nell’attuazione della politica agricola comune, ha fatto anche una scelta politica: tra le misure nazionali

condividiamo tutte le considerazioni che sono state fatte, si può dire che sul tema dell’efficienza delle strutture irrigue, dell’efficienza energetica e sull’utilizzo proficuo delle risorse idriche

ben oltre dodici anni. Non era più una gestione commissariale, ma una gestione che andava normalizzata e che oggi rientra nelle piene attività del Governo

individuata anche una misura nazionale nel programma nazionale di sviluppo rurale: oltre alle risorse che vengono messe a disposizione dalle Regioni, c’è una misura nazionale per l’intervento sulle infrastrutture irrigue.

in tale contesto ben si comprende la crescente richiesta da parte dei consorzi meridionali di assistenza e supporto tecnico, cui le Regioni competenti dovrebbero dare puntuale riscontro, avvalendosi, eventualmente, anche dell’assistenza tecnica assicurata nell’ambito dei Programmi di sviluppo rurale;

riguardanti le infrastrutture irrigue del Meridione e gli impianti idroelettrici finanziati, mediante l’adozione di ogni opportuna iniziativa tesa a salvaguardare le attività opportunamente poste in essere prima dalla struttura tecnica commissariale e successivamente dai competenti dipartimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

«Ad assumere le opportune inizia-_ tive, volte ad assicurare agli enti attuatori, le condizioni minime per realizzare al meglio le infrastrutture necessarie agli interventi idrici e irrigui». Su questo punto il parere è favorevole «nei limiti delle competenze statali».

a livello locale; 5) a valutare la possibilità di elaborare, d’intesa con le Regioni, un piano per la realizzazione di piccoli invasi gestiti da consorzi di agricoltori

in tutta sincerità, mi pare un po’ incredibile che si possa dire che non si devono realizzare le opere che già risultano iniziate.

Signora Presidente, colleghi, le mozioni presentate quest’oggi rappresentano un’occasione per discutere in merito all’annoso problema dell’inadeguatezza delle infrastrutture irrigue nel nostro Paese. In questo contesto, gli elementi critici che dobbiamo prendere in considerazione sono: da una parte, la tutela dell’acqua, come bene naturale e diritto universale dell’essere umano; dall’altra, l’utilizzo dell’acqua quale risorsa necessaria e indispensabile per garantire l’esistenza ad ogni essere vivente, in primis al genere umano. In merito al primo punto, è evidente che l’acqua è un bene «finito», quindi dobbiamo garantire alle future generazioni la sua disponibilità ed evitare di alterare gli ecosistemi esistenti. Per ciò che concerne il secondo punto, invece, è necessario trovare delle modalità attraverso cui l’uomo moderno non debba rinunciare alla vita a cui l’economia globale ci ha abituato. Lo sviluppo tecnologico moderno ormai ci consente di adottare un modello di sviluppo sostenibile applicato al sistema al sistema agricolo, senza alterare l’ambiente e compromettere gli habitat naturali. Ciononostante, ci troviamo a gestire una situazione emergenziale.

Nello stesso periodo la Regione Puglia, per fare un esempio, è arrivava a disperdere la metà dell’acqua condotta. A questo contesto va sommato l’effetto di eventi climalteranti (siccità, alluvioni, piogge torrenziali)

gli attuali consorzi di bonifica, che dovrebbero provvedere alla redazione delle progettazioni e alla realizzazione delle opere, non si sono dimostrati all’altezza dei compiti loro assegnati. La conseguenza è che ci troviamo a dover gestire una serie di lavori iniziati e non terminati. Ciò vuol dire che il progresso tecnologico da solo non può sostituirsi alle scelte politiche,

e coinvolge i due terzi della disponibilità mondiale di acqua dolce, appare chiaro che la necessità di intervenire è divenuta improcrastinabile. Per quanto riguarda la riduzione dei consumi, il riutilizzo delle acque reflue depurate è uno dei fattori d’intervento più importanti. Se la qualità dell’acqua recuperata è opportunamente gestita, le acque reflue trattate possono fornire un’alternativa efficace per soddisfare la domanda d’acqua dell’agricoltura, soprattutto quando si verificano fenomeni di siccità o di carenza di risorse idriche. Il vantaggio del riutilizzo risiede, infatti, nella possibilità di fornire un approvvigionamento idrico alternativo, valido almeno per gli usi che non richiedono acqua di elevata qualità, che può ridurre il consumo delle acque sotterranee. Basti pensare che nel 2000 a causa della siccità la sola agricoltura pugliese ha subìto danni per 836 milioni di euro. Dobbiamo recuperare il tempo perso. È quindi auspicabile che il Governo, di concerto con le Regioni ed i Comuni, metta in atto un piano nazionale per uscire dall’emergenza, principalmente potenziando le risorse finanziarie e sbloccando quelle che già sono state destinate a questi interventi,

che determinano l’aumento costante della temperatura media globale del pianeta, di cui si è occupata la COP21 a Parigi lo scorso anno e di cui si occuperà

del nostro Paese. La cancellazione dell’Agensud, che apparteneva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’introduzione di un commissario ad acta, dopo la cancellazione dell’Agensud, il passaggio di competenze dal commissario ai diversi dipartimenti del Ministero delle politiche agricole purtroppo non hanno accelerato, come la gente auspicava, l’attività connessa all’attuazione del programma irriguo nazionale. Nel nostro Paese, soprattutto nel Meridione, le reti irrigue e le infrastrutture idriche sono assenti o sono vecchie. Laddove esistono sono inefficienti, perché non viene fatta manutenzione. Esistono elevate perdite di acqua, con conseguenti costi enormi per i cittadini. Tutto questo non è un caso. Certamente ci sono i cambiamenti climatici. Ma questo è legato soprattutto a una gestione dissennata dei consorzi di politica, inefficienti ed inefficaci,

profumate sanzioni europee. Pensiamo, per esempio, allo scandalo della gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia, dove - è paradossale - non esiste ancora un piano regionale regionale dei rifiuti. Invece che basarsi su impianti di trattamento, lì si lavora ancora e si smaltisce facendo ricorso alle discariche. Detto questo, il Gruppo della Lega Nord condivide sostanzialmente le tre

in corso riguardante infrastrutture irrigue e impianti idroelettrici già finanziati. Ci sta bene valutare progetti di investimenti congrui che perseguono soprattutto - questo è un tema che ha sottolineato il collega Piccoli - l’efficientamento energetico fino all’autosufficienza. Ci sta bene avviare una seria riflessione e discussione sui sistemi di consorzi di bonifica, Ci piacerebbe che, dopo l’approvazione di queste mozioni, ci fosse un impegno periodico da parte del Governo che, delegando le Commissioni

sulla necessità di una pianificazione attenta delle risorse idriche del nostro Paese, le quali rappresentano un patrimonio vitale vitale per lo sviluppo, su cui impattano, però - su questo forse dovevamo concentrarci di più - in modo imponente ormai i fenomeni di cambiamento climatico, come l’innalzamento delle temperature.

le famose bombe d’acqua. È chiaro che, soprattutto per il settore agricolo, affrontare con serietà la questione della gestione delle risorse idriche diventa vitale per la sopravvivenza stessa dell’agricoltura, così come è vitale per la difesa del suolo. 2016 Innanzitutto, dovremmo mettere a regime un piano per il risparmio idrico, quindi per una gestione razionale delle risorse contro gli sprechi. Contemporaneamente, però, abbiamo necessità di una gestione adeguata della rete infrastrutturale, che assicuri il mantenimento e la funzionalità. È pertanto assolutamente necessario e urgente

infatti, che il Ministero ha il compito di garantire che il passaggio delle competenze da Agensud all’ente commissariale non debba tradursi in ulteriori rallentamenti;

pure che, rispetto al superamento dell’ex Agensud, da parte del Ministero erano state trasferite una serie di di funzioni e assegnati specifici compiti aggiuntivi in materia di razionalizzazione. Quindi, onestamente, non capiamo la necessità di un ulteriore rafforzamento della gestione commissariale, soppressa più di un anno fa, perché tutti gli impegni del testo di questa mozione, connessi al presupposto della salvaguardia delle attività poste in essere dalla struttura commissariale, francamente non ci sembrano molto positivi. positivi. Torniamo a ripetere che le azioni di cui necessita il settore delle infrastrutture vanno viste in un’ottica sistemica, valorizzando il livello locale, risistemando la questione dei consorzi di bonifica e soprattutto facendo in modo che i finanziamenti per il Piano irriguo nazionale si parla di 800 milioni nel periodo di programmazione 2014-2020 - siano ben utilizzati. Tra l’altro, il CIPE ha assegnato più di 400 milioni di euro dei fondi al settore dell’agricoltura

Abbiamo sentito dire che ci sono problemi connessi ai cambiamenti climatici, cosa sacrosanta, verissima e sotto gli occhi di tutti. Un problema più grave con cui dobbiamo confrontarci è, purtroppo, l’intensa urbanizzazione del suolo, perché il problema della bonifica deriva non solo dall’incremento di precipitazioni concentrate in un tempo molto stretto, ma anche da una diminuzione del coefficiente di assorbimento del suolo.

abbiamo anche incrementato in maniera molto forte le superfici coltivate a serra. Anche questo ha prodotto un notevole incremento del coefficiente di deflusso nei corsi d’acqua naturali e artificiali. Quindi, ci troviamo di fronte a una situazione del suolo completamente cambiata. I consorzi avevano il ruolo di garantire la bonifica e di evitare gli allagamenti dovuti a questo forte incremento delle acque scolanti,

c’è una confusione incredibile. Ciò che dovrebbe fare uno Stato serio è rimettere in ordine le competenze. Questo dovreste fare e questo è quello che ci auguriamo che voi facciate.

intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia alle tre mozioni presentate, con la sottolineatura che crediamo che questo

Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l’ordine di presentazione. Passiamo alla votazione della mozione

Signora Presidente, signora Sottosegretario, ono- revoli colleghi, la legge quadro n. 394 del 6 dicembre del 1991 sulle aree protette sta per compiere e, dopo tutto questo tempo, possiamo affermare che è stata una buona legge; una legge nata grazie all’importante lavoro svolto, alla fine degli anni Ottanta, dalle associazione ambientaliste e alla capacità di ascolto della politica e delle istituzioni, che ha aperto la strada alla stagione dei parchi nel nostro Paese. È bene ricordare, colleghi, che le aree protette nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati del 2010, sono 871, per una superficie protetta a terra di 32.000

Parliamo complessivamente di 24 parchi nazionali, 29 aree marine protette e 152 parchi regionali. Nel frattempo, dal 1991 a oggi, il contesto in cui si inseriva la legge quadro è significativamente cambiato; ad esempio, è mutato l’assetto istituzionale nel nostro Paese, sono state introdotte nuove normative a livello europeo nel campo della conservazione e della tutela dei beni naturali; è cresciuta l’attenzione e la consapevolezza… (Brusio).

degli effetti del climate change e della relativa ne- cessità di tutelare la biodiversità. Per questi motivi, una modifica della legge è necessaria. Non dobbiamo aver paura di aggiornare una normativa che risente del tempo e che necessita di una versione 2.0, per il rilancio dell’attività delle aree protette e la gestione delle nuove competenze che vogliamo attribuire Colleghi, superare gli scetticismi è difficile: sappiamo bene quanto sia più semplice creare consenso per il mantenimento dello status quo. Ma la scommessa che ci attende oggi non è difendere l’esistenza dei parchi - a cui nessuno sta attentando bensì creare le condizioni affinché essi assolvano al meglio alle proprie funzioni: tutela e accrescimento della biodiversità; promozione di buone pratiche nell’uso delle risorse naturali; educazione alla sostenibilità e valorizzazione dei territori e delle economie locali. Il sistema delle aree protette tocca, con intensità differenti, oltre la metà dei Comuni italiani, costituendo un’importante risorsa verde anche per le grandi città. A mio parere i parchi, come prezioso strumento di gestione delle risorse naturali e del territorio, o vivono ed espandono la propria attività di motore dello sviluppo sostenibile fuori dai propri confini, dialogando quindi con le realtà territoriali su cui insistono, oppure sopravvivono nell’inutilità, nell’autoreferenzialità o, peggio ancora, possono trasformarsi nella foglia di fico dietro cui nascondere i vari atti di aggressione al territorio e al paesaggio perpetrati da amministratori poco avveduti o da imprenditori spregiudicati. I parchi devono essere vissuti come uno strumento utile, vicino alle persone, in grado di migliorare le nostre condizioni di vita, strumenti virtuosi di politiche pubbliche capaci di sollecitare l’azione dei soggetti privati disposti a scommettere sull’economia verde.

vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per portare il provvedimento fin qui: il Presidente e tutti i colleghi della Commissione ambiente, il consigliere De Salvo e i funzionari della Commissione, la Direzione aree protette e l’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente. L’iter in Commissione di questo disegno di legge è stato molto lungo proprio perché eravamo consapevoli della difficoltà di agire su una legge così importante. L’attività istruttoria, checché se ne dica, è stata particolarmente approfondita. Abbiamo proceduto ad un’articolata fase di ascolto di tutti i portatori di interesse delle aree protette. Venticinque è il numero di audizioni svolte in Commissione, tra cui quelle delle più rappresentative associazioni ambientaliste, senza contare le missioni nei territori dei vari parchi. Abbiamo svolto trentasei sedute in sede referente. Al Testo unico sono stati presentati un totale di 1.884 proposte emendative: un lavoro di sintesi importante che ci ha portati al testo che ci apprestiamo a discutere, un testo che basa il suo impianto su una governance più snella e rafforzata per le aree protette. Il problema dei lun- ghi commissariamenti e delle mancate intese viene eliminato, diventa più forte il ruolo del Presidente del parco, sempre nominato con decreto dal Ministero dell’ambiente previa intesa della Regione o delle Regioni sul cui territorio ricade l’area protetta, nell’ambito di una terna di soggetti con una comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni e nella gestione di strutture pubbliche o private. La carica diventa incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

sentite le Commissioni parlamentari competenti - badate bene - scegliendo prioritariamente tra i nomi della terna e non, come ho sentito dire, discrezionalmente tra gli uomini di fiducia del Ministro. Colleghi, permettetemi un inciso: non credo che i Presidenti dei parchi debbano connotarsi solo per l’ottimo curriculum scientifico, devono bensì possedere l’esperienza e la capacità per sapersi misurare con i contesti di riferimento, così come i direttori che invece di assurgere al ruolo di dirigenti ministeriali, che decidono da soli cosa è meglio fare, diventano lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi che gli organismi preposti - il presidente, il consiglio del parco e la comunità del parco - definiscono. Non basta che le nomine siano fatte da istituzioni il più distanti possibile dal territorio dove insiste il parco per avere la garanzia della loro qualità. La nomina di un direttore, fatta in maniera discrezionale da un Ministro, non può essere migliore di quella fatta da un buon consiglio direttivo. Con l’abrogazione dell’albo dei direttori di parco prevediamo, quindi, una nuova e più trasparente procedura per la nomina del direttore che sarà designato dal consiglio direttivo sulla base di una terna. La terna sarà il risultato di una selezione pubblica tra profili di comprovata esperienza nella gestione delle aree protette e dell’amministrazione pubblica. Cosa vuol dire? Mentre ora abbiamo un albo composto principalmente da uomini e donne (poche) sopra i cinquant’anni, alcuni dei quali addirittura senza laurea, d’ora in poi solo i vincitori di concorso con 3 Novembre 2016 nale nelle aree protette, sia terrestri che marine, potranno ambire a questo importante ruolo. Abbiamo modificato la composizione del consiglio direttivo, che avrà dai sei agli otto membri e sarà designato per il 50 per cento dalla comunità del parco. Tutto questo per risparmiare tempo e denaro, e rendere le decisioni più rapide e agevoli in capo a un presidente a più diretto contatto con la comunità del parco, sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e dei revisori dei conti. L’obiettivo è chiaro. Avvicinare il parco al territorio, senza che questo perda il contatto con un sistema nazionale e internazionale di conservazione della natura. I parchi non sono il fine della conservazione, ma uno dei mezzi, seppur fondamentale, per raggiungere le nuove frontiere della conservazione. I parchi, quando sono isolati, anche quelli meglio gestiti, non raggiungono quasi mai significativi risultati nella conservazione degli habitat, specie se non sono inseriti all’interno di una rete ecologica e se non sono guidati da una strategia nazionale per la conservazione della biodiversità. Abbiamo voluto riproporre un nuovo comitato per le aree protette

finalmente tutte le aree protette del nostro Paese, e per definire gli obiettivi e le azioni da compiere per raggiungere gli obiettivi nazionali e sovranazionali di tutela della biodiversità. A rafforzare ancora di più il sistema nazionale delle aree protette abbiamo inserito nel testo una grande novità: le aree del territorio inserite nella rete ecologica europea definita Natura 2000, SIC e ZPS, ricadenti interamente o parzialmente, e addirittura quelle esterne all’area protetta, saranno gestite dal parco e concorreranno, assieme ad esso, alla conservazione della biodiversità. Inoltre, laddove esistano delle aree marine protette che confinano con un parco terrestre si va a formare un ente unico, classificato come parco nazionale con estensione a mare. Altro capitolo importante è il piano del parco. Mantenendo le finalità fondamentali di tutela dei valori naturalistico-ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali, il piano del parco assorbe il piano economicosociale, che viene abrogato, e assume anche il ruolo di strumento con il quale il parco può disciplinare iniziative economiche di valorizzazione del territorio del patrimonio edilizio tradizionale e agro-silvo-pastorali nonché di turismo sostenibile. Al piano, il cui iter di approvazione viene semplificato, viene rico- nosciuta anche la valenza paesaggistica (e questo è un altro aspetto molto importante), rafforzata dall’obbligo di valutazione ambientale strategica. 2016 semplificare le procedure del codice urbano, che dal 2004 prevedeva la doppia autorizzazione, dell’ente parco e della sovraintendenza, anche per interventi di modesta entità, è previsto, in vigenza del piano con valenza paesaggistica o in assenza del piano

Attraverso il piano, il parco può inoltre definire le aree contigue di intesa con la Regione. Nelle aree contigue il parco il parco regolamenta l’attività venatoria ed estrattiva e la pesca. Sempre nel piano del parco si definiscono gli obiettivi di conservazione specifici per ogni area protetta. controllo della fauna selvatica, viene introdotto il divieto esplicito di caccia nei parchi. Per la salvaguardia della biodiversità vengono introdotti piani di gestione della fauna selvatica di competenza dell’ente parco con il parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA e l’impiego di personale qualificato, dipendente o esterno, ma con formazione certificata dall’ISPRA stessa. I piani prevedono il contenimento - a partire dai metodi non cruenti fino alla cattura e, solo come ultima istanza, all’abbattimento, sempre con il parere vincolante dell’ISPRA delle specie che possono comportare danno alla biodiversità e rischi per l’incolumità umana. Per quanto concerne servizi ecosistemici e royalty, i gestori di im- pianti elettrici, attività estrattive, impianti a biomasse, coltivazioni di idrocarburi, oleodotti, metanodotti, elettrodotti non interrati e pontili di ormeggio per imbarcazioni, già presenti e attivi all’interno dei parchi al momento dell’entrata in vigore della legge, dovranno corrispondere un contributo agli enti per i servizi ecosistemici offerti. Una parte cospicua di questo contributo confluirà in un fondo, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinato al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell’area parco. I parchi avranno inoltre la facoltà di imporre ai visitatori un ticket per i servizi offerti e di concedere a titolo oneroso il proprio marchio, di stipulare contratti di sponsorizzazione, di disporre dei beni demaniali e di quelli confiscati alle mafie. Al Governo viene affidata una delega per l’introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici offerti dalle aree protette, come era stato previsto nella legge sulla green economy, il famoso collegato ambientale. Poi c’è la partita dei nuovi parchi:

area protetta marina e parco terrestre. C’è poi la grande scommessa dal Parco del delta del Po, parco interregionale, con una delega al Governo per la sua istituzione. L’area deltizia più importante d’Europa muove da una situazione di stallo, si dà la possibilità di realizzare un parco interregionale, con una regia unica, prodromico alla nascita di un parco nazionale. Credo sia un passo importante e significativo che bisogna saper cogliere nella sua importanza per proseguire poi Con questo provvedimento, come dicevo poc’anzi, abbiamo anche rimediato a ferite e dimenticanze della

per la prima volta l’ISPRA avrà una parola importante nella definizione della strategia di conservazione dei nostri ecosistemi e dei parchi. A ogni parco è stato dato, all’interno del Piano del parco, un obiettivo in termini di conservazione da raggiungere, che deve essere rendicontato annualmente, tramite il Comitato per le aree protette, al Parlamento: quindi, il massimo del

la promozione dei parchi in Italia e una pietra miliare della conservazione di questo Paese. Mi avvio alla conclusione: di legge vuole riaccendere l’interesse delle istituzioni verso i parchi con l’intento di ricondurli nel più ampio quadro delle strategie mondiali e comunitarie per la conservazione della biodiversità per arrestarne la perdita, facendo in modo che anche i parchi siano parte attiva per la lotta ai cambiamenti climatici e al mutamento degli habitat. Con questa proposta noi riteniamo di aver dotato i parchi di qualche strumento in più per mettersi al servizio delle comunità e per contribuire al miglioramento del Paese. Concludo, cari colleghi, ricordando un aspetto per me molto importante e anche emozionante. Nel mio percorso di ascolto, che ha toccato gran parte della penisola, quale ancora una volta ho potuto apprezzare le bellezze straordinarie del nostro Paese, dal Nord al Sud, passando per il Centro e le nostre stupende isole, grazie al collega

quella legata in maniera indissolubile a Norcia e a Castelluccio. Ebbene, a Ussita, io e il collega Morgoni, in un’affollata assemblea pubblica, abbiamo incontrato semplici cittadini, imprenditori, pastori, allevatori e operatori turistici, soprattutto giovani e donne,

decisamente alle opportunità straordinarie che il parco offriva loro; con protagonismo hanno accorciato le distanze che molte volte si palesano tra le decisioni romane e le priorità rappresentate dalle comunità locali.

senza dimenticare Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e le centinaia di borghi del nostro entroterra colpiti più volte e in maniera drammatica dal terremoto. Lavoriamo, colleghi, affinché possano tornare al più presto nei luoghi di appartenenza alle loro attività, a fare comunità. Il parco deve diventare protagonista e vettore della buona ricostruzione, della memoria, del buon uso del territorio; si deve poter vivere e trarre benefici, non solo di natura economica, ma anche in termini di qualità della vita in questa straordinaria e bellissima montagna. I Monti Sibillini, con il loro parco, devono diventare il paradigma di un’Italia che vuole valorizzare la bellezza del paesaggio e difendere un ecosistema dove le persone vivono bene, con grande afflato con la natura. A tutti loro dobbiamo tendere in uno straordinario sforzo comune, a tutti loro dobbiamo offrire non solo la nostra solidarietà, il nostro abbraccio e la nostra vicinanza, ma anche dare dimostrazione di capacità politica,

nuovi elementi istitutivi che possano effettivamente monitorare il lavoro che viene svolto all’interno dei parchi e il livello di qualità della gover_nance dei parchi stessi._

come un vincolo, ma non come quell’opportunità economica e premiale per territori di particolare pregio. Ancora, sono mancati alcuni strumenti economici ed operativi

la possibilità di venire finanziati per migliorare la conservazione, renderla fruibile e rendere possibile e migliorabile quel turismo ecologico che oggi è in crescita esponenziale e che può garantire molto lavoro a figure specialistiche, soprattutto ai giovani. Dunque cambiare per migliorare: questo era per noi importante, ma non facile. Mesi di lavoro, tantissime audizioni un’enormità di emendamenti hanno portato a questo risultato, e altri probabilmente ne vedremo nel corso del dibattito in quest’Aula. Passo ad identificare gli elementi caratteristici, a mio avviso, delle modifiche inserite. Come detto, vi sono nuove modalità manageriali e nuove modalità di finanziamento, che contribuiranno ad ad attuare il riconoscimento dei servizi ecosistemici, e dunque a riconoscere il valore della gestione e del mantenimento di quel capitale naturale che abbiamo la fortuna di avere. Cito per titoli. Dal contributo di sbarco a favore delle isole minori per le aree protette all’inserimento degli enti parco tra i beneficiari del cinque per mille della legge sull’IRPEF del 2006: dopo università, ricerca scientifica e volontariato, avremo anche gli enti parco che potranno beneficiare di questo importante cinque per mille. degli incassi degli enti parco nazionali verrà depositato in un fondo per implementare interventi che favoriscano biodiversità, habitat naturali, finanziamenti di progetti e azioni di sistema. Qualsiasi attività ambientale già esistente o in qualche modo insediabile, naturalmente previa verifica, all’interno degli stessi parchi italiani dovrà inoltre versare una royalty speciale ai gestori del parco, con un doppio significato: quello di contribuire alla valorizzazione, ma anche come atto risarcitorio, per contribuire agli effetti di mitigazione necessari e per dare valore alla specificità di un ambiente fragile e da proteggere. Penso ancora a quella quota per il momento minima, ma che vorremmo incrementare, relativa al fondo per gli abbattimenti degli animali non autoctoni, che verrà utilizzato per la ricerca di metodi di gestione non violenti e non cruenti di una fauna selvatica impropria.

un’altra questione importante ed è la seconda che voglio rilevare: niente più approssimazione e conflitti di competenze scientifiche o tecniche relativamente agli interventi necessari a garantire la corretta gestione dei parchi. L’ISPRA - è stato detto - assume con questa legge un ruolo di enorme rilevanza, garantendo tutti - tutti davvero - nessuno escluso. L’ISPRA è dunque chiamato al supporto scientifico-tecnico, al monitoraggio, al controllo ambientale e dovrà occuparsi anche di individuare gli strumenti operativi di piano per i piani di eradicazione o limitazione di specie alloctone e per valutare la modalità di intervento di qualunque genere nelle aree protette; concetto, come si è detto, ampliato alle zone a protezione speciale ai siti di importanza comunitaria e alle zone speciali di conservazione. Abbiamo eliminato la caccia selettiva dentro i parchi, che era prevista come eccezione purtroppo non vedeva un divieto esplicito nella normativa attualmente esistente. Cambiano anche le modalità con cui si regolamentano i rapporti tra gli enti parco e i Comuni relativamente alla gestione dei piani. Cambiano i rapporti tra le Regioni relativamente alle nomine. Quindi si estendono e si applicano i regolamenti per l’adeguata gestione dei parchi e delle aree marine protette con tempi certi e responsabilità chiare.

pronuncia o nulla osta da parte della pubblica amministrazione verso i gestori dei parchi debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta intendendosi altrimenti favorevole; dunque certezza nelle nomine nei consigli di amministrazione e nei direttori degli enti parco. Lasciatemi citare il caso vergognoso della presidenza del Parco delle Dolomiti, mai nominata da un anno e mezzo per conflitti perenni tra Stato e Regione, con una vacanza amministrativa e gestionale che ha già ha ritardato e ritarderà la realizzazione di progetti e farà perdere finanziamenti europei. Quindi, basta a tutto questo. Mi

dell’istituzione di un parco interregionale in quest’area, è una ciliegia sulla torta in questa riforma delle aree a parco italiane. Un provvedimento che vedrà la luce in accordo con le due Regioni e le comunità locali, ma finalmente vedrà questa zona umida, di straordinario valore, prospiciente il mare Adriatico e con una realtà faunistica di incredibile ricchezza nel suo genere - definita, non a caso, la Camargue italiana, ma molto più estesa e, lasciatemelo dire, molto più bella - tentare la via di una governance capace di valorizzare a scopi di tutela, salvaguardia e promozione turistica, un patrimonio comune di straordinaria bellezza. Gestione fluviale, costiera, recupero per altri scopi di attività industriali dismesse; fino a poco fa pensavamo - pensate quanto siamo assolutamente stupidi - di reinvestire nella centrale di Porto Tolle. Tutto questo diventerà invece piano per sviluppare da parte dell’ente gestore del Parco, in collegamento con le comunità locali,

quella che possiamo mettere in campo, anche grazie a questo provvedimento, verso il mantenimento di quella bellezza di cui godiamo troppo spesso inconsapevoli, ma anche ai fini di una corretta governance e ai fini di quel necessario sviluppo compatibile, in punta di piedi, ma con enorme portata e rilevanza economica, sociale, ambientale e di lavoro. (Ap- Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, volevo ricordare che per questo disegno di legge l’11 settembre 2013, oltre tre anni fa, venne votata la procedura di urgenza per procedere all’esame abbreviato dello stesso, ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento del Senato. 3 novembre 2016; sono passati oltre tre anni e questo certamente non è per colpa del bicameralismo paritario. premessa. La Lega Nord ha sempre ritenuto importante, per la stessa conservazione della specie umana, il contrasto della tendenza alla perdita della biodiversità attraverso la tutela delle aree protette e degli ecosistemi. Studi scientifici dimostrano come la stabilità degli ecosistemi incida anche sulla salute umana. Il nostro Paese detiene il primato europeo della biodiversità; ha una dotazione importante di habitat, molti di questi dichiarati prioritari a livello comunitario. Tra parchi nazionali e regionali e aree marine protette risulta protetto circa il 12,5 per cento del territorio nazionale, una percentuale che, sommata alle aree protette a livello europeo, ossia ai siti di interesse comunitario (SIC) e alle zone di protezione speciale, arriva persino al 21,8 per cento. Queste percentuali sono in continuo aumento. Si tratta di una ricchezza che occorre valorizzare adeguatamente quale risorsa vera e propria del nostro territorio e da non trattare come un mero vincolo territoriale. Secondo il nostro Gruppo, le Regioni e gli enti locali, ossia le istituzioni più vicine alle necessità del territorio e dei cittadini, devono essere i soggetti responsabili della governance delle aree protette e della copianificazione paesaggistica. Il permanere delle aree protette nazionali risponde ormai a esigenze di mero finanziamento delle spese correnti degli enti parco vista l’esiguità delle risorse disponibili, interessa solo quelli meno virtuosi che non sono in grado di sviluppare finanziamenti mediante idonee pratiche di autofinanziamento, di sviluppo del turismo sostenibile e di promozione dei prodotti tipici. Una delle riforme importanti proposte dal disegno di legge è la semplificazione per l’istituzione delle aree marine protette prevedendo l’estensione dei parchi nazionali terrestri anche nelle aree protette marine contigue. Purtroppo, però, non si prevede la possibilità di istituire aree marine protette e riserve marine anche da parte delle Regioni al fine di evitare, per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali, una doppia gestione con oneri con oneri a gravare sulle finanze pubbliche. Riteniamo tale carenza molto grave, dal momento che il sistema delle aree marine protette è in sofferenza a causa delle ridotte disponibilità finanziarie per la gestione ordinaria e per gli investimenti. Anzi, l’istituzione di riserve marine in corrispondenza di tratti di costa dove sono già presenti enti gestori di aree protette regionali dovrebbe essere prioritaria nell’ambito della riforma. Un altro concetto non condivisibile è l’individuazione di un territorio contiguo nell’area del parco che, nonostante sia esterno al perimetro del parco, viene sottoposto alla governance dell’ente parco stesso. Non riteniamo opportuno che il regolamento del parco definisca l’esercizio delle attività anche nelle aree ad esso contigue e nelle aree SIC e nelle zone di protezione speciale, che anche parzialmente ricadono nel perimetro del parco, sottraendo con ciò

possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive per la tutela dell’ambiente. Se si pensa alla grande estensione del territorio protetto nazionale in continuo aumento, si tratta di un’imposizione di divieti assurdi che non rientrano nella giurisdizione dell’ente parco. Un’altra grande novità introdotta con il presente disegno di legge è l’imposizione di addizionali a tutti i canoni concessori alle concessioni idroelettriche, alle attività estrattive, al passaggio di oleodotti e metanodotti, e metanodotti, ai beni demaniali, a titolo di contributo alle spese dell’ente parco per il recupero della naturalità. Senz’altro lo scopo è quello di trovare finanziamenti per la gestione dei parchi, vista la penuria delle risorse statali. Peraltro, tale imposizione non riguarda solo le aree interne al perimetro del parco - anche perché alcune attività sono proprio vietate all’interno dei parchi - ma riguarda anche tutte le aree contigue. Sono sottoposti alla nuova tassa anche gli agricoltori titolari di impianti a biomassa nelle aree del parco e nelle aree contigue: si tratta di una tassazione, per noi della Lega Nord, inaccettabile. Non si capisce poi il perché dell’esonero dal contributo per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti già in esercizio nei parchi. Parliamo dell’eolico e del fotovoltaico, impianti veramente impattanti, comunque più degli oleodotti e metanodotti. in ogni caso, di un innalzamento della tassazione che non si ritiene condivisibile, specialmente nel periodo di crisi economica attuale e in considerazione delle difficoltà che le nostre imprese della tanto pubblicizzata dal Governo semplificazione e razionalizzazione delle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi? Da una parte, Governo e maggioranza semplificano le disposizioni della Conferenza di servizi contenute nella legge n. 241 del 1990, come modificata successivamente, prevedendo forme di raccordo tra le amministra a pronunciarsi sulle autorizzazioni di interesse per le imprese, comprese quelle ambientali, introducendo meccanismi diretti a superare situazioni di inerzia; dall’altra parte, invece, nel presente provvedimento, eliminano il silenzio-assenso sull’inerzia del parco nell’esprimere il parere sugli interventi infrastrutturali, anche per i casi di interventi edilizi minori, ove l’autorità competente al rilascio dei permessi di costruire o lo stesso professionista abilitato sarebbero già in grado di controllarne la compatibilità con il regolamento Riteniamo che l’inerzia colpevole dell’ente parco non dovrebbe e non debba determinare la paralisi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione. Un’altra questione da segnalare è l’eliminazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle aree contigue del parco. Non si comprende la ratio della norma dal momento che il disegno di legge estende la governan- il regolamento del parco anche alle aree contigue, ma restringe la pos- sibilità degli indennizzi nell’area del parco, eliminando peraltro i risarcimenti che potrebbero risultare più onerosi per gli enti parco ma meno accettabili per i cittadini danneggiati. Si condivide la diminuzione degli organi degli enti parco attraverso l’eliminazione della giunta, la diminuzione dei membri del consiglio direttivo e dei revisori, l’eliminazione del comitato d’esame per i pareri su concessioni autorizzazioni, ma non si condivide il previsto silenzio-assenso sull’intesa con la Regione per la nomina del presidente dell’ente parco. Inoltre, l’assenza dell’intesa con la Regione per la nomina dei consiglieri

mette in osservazione della fase della trattazione degli emendamenti, a questo punto rinviata alla prossima settimana, per una valutazione e per le considerazioni più opportune che porteranno all’espressione del voto finale del nostro Gruppo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut.

che chiaramente ripercorre quanto riportato in questo disegno di legge, è a mio

Il senatore Caleo ha dato una visione assolutamente non reale di come oggi stanno le cose.

che, all’interno del Parco, sono l’espressione dei cittadini. Attraverso la loro volontà democratica si esprimano e si tenga assolutamente conto della volontà delle genti che abitano all’interno dell’area Parco del Delta del Po.

Piccoli). PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze e considerando che molti colleghi ritenevano che il dibattito precedente si sarebbe prolungato, ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

il mondo del lavoro è peggiorato totalmente. La disoccupazione sale ancora e purtroppo è arrivata ad un picco dell’11,7 per cento. Prima se ne va questo signore e meglio è per tutti gli italiani.

occorre fronteggiare l’emergenza delle persone e l’inagibilità delle case. La moltitudine di sfollati ovviamente allarma e richiede l’attenzione di tutti. case c’è un altro aspetto da tenere in considerazione. Mi riferisco a tutte le grandi infrastrutture, come ponti, tunnel, opere idrauliche. In particolare, in Provincia di Macerata, nel Comune di Cingoli, c’è un lago, il lago artificiale di Castreccioni, con una diga e un viadotto che vengono considerati ad alto rischio

o si interviene tempestivamente per accertare l’effettiva pericolosità, e quindi si mette in sicurezza il viadotto, o noi, signori miei, rischiamo potenzialmente un secondo Vajont. Vajont. Siccome siamo sempre soliti piangere dopo che le cose accadono e non prima, spererei che in questo momento, visto che la terra trema di suo,

in questi ultimi giorni la Calabria dell’istruzione negata, del diritto alla scuola etereo e metafisico, grazie a quanto ci ha fatto sapere «Report», «Report», sta vivendo un altro dramma in un piccolo paese: Serra d’Aiello. È un dramma che impedisce a 16 bambini della scuola primaria di poter esercitare il diritto Questi ragazzini, a causa di problemi - di cui la prefettura stessa è a conoscenza - insorti tra le amministrazioni comunali di Serra d’Aiello e di Amantea, e di Amantea, non riescono a sfruttare, come è nel loro diritto, un trasporto scolastico pubblico gratuito. Pertanto, a questi 16 bambini viene negata la possibilità di non diventare NEET, di non diventare manovalanza per la criminalità organizzata, di non diventare bacino potenziale per tutti quei fenomeni di devianza e perversione per cui, alla fine, noi ci indigniamo. Se uno Stato vuole investire in istruzione e cultura attraverso gli enti territoriali deve far fronte a queste emergenze. L’anno scolastico è cominciato da tanto, tanto tempo. Aggiungo un ultimo un ultimo dato di riflessione. Serra d’Aiello vanta 450 residenti. Negare la possibilità di frequentare la scuola a 16 bambini in età di scuola primaria è un assoluto crimine. Guarda caso, a Serra d’Aiello si pensa però di investire tanto denaro pubblico perché si vuol realizzare - così si apprende da fonti di stampa - un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e, addirittura, di 450 residenti, si prevede l’arrivo di forse anche 1.000 extracomunitari e richiedenti asilo. Sulla struttura in questione, che un tempo ha occupato tanto spazio sui giornali locali e che è stata definita una struttura lager (perché purtroppo ci sono stati anche casi di cronaca nera),

un collega che come lui conosce professionalmente le dinamiche e il funzionamento del mercato del lavoro si accodi, in modo così fazioso e apparentemente ingenuo, alla falsificazione - perché di questo si tratta - diffusa nell’informazione quotidiana

rispetto al periodo corrispondente del biennio 2013-2014, ci sono state complessivamente 1.214.662 assunzioni in più. Di queste, più di due terzi (818.306) a tempo determinato ed un terzo (396.356) a termine. Questo è il dato. E questo significa che se in aumento, la disoccupazione aumenti di un punto decimale, ciò è dovuto soltanto al fatto che dei lavoratori prima inattivi entrano in un mercato del lavoro in cui riacquistano la speranza di trovare un’occupazione. Ma sia in termini di stock (cioè di livello complessivo di occupazione, dove abbiamo circa 700.000 posti di lavoro in più, di cui due terzi a tempo indeterminato nell’ultimo biennio), sia in termini di flusso il segno è nettamente positivo. Questo ho ritenuto di dover precisare perché in quest’Aula, almeno qualche volta, si dicano le cose vere e vengano corretti i dati falsi su

Signora Presidente, intervengo perché ho ap- preso solo adesso cosa sta accadendo a Catania. In un quartiere della mia città, i negozi hanno dovuto chiudere le saracinesche tutto il giorno perché oggi, alle ore 16, si celebrerà il funerale del figlio di un pregiudicato. ho richiesto l’intervento del prefetto e delle Forze di polizia affinché Catania non diventi il palcoscenico di un’esibizione di potere mafioso.